Pertanto, come già preannunciato nella seduta di martedì 11 gennaio, domani, alle ore 9, si svolgerà la relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia. Al termine della seduta il Senato sarà convocato a domicilio. Lunedì 24 gennaio, alle ore 15, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sempre lunedì 24 gennaio, rispettivamente alle ore 10 e alle ore 12, sono convocate le riunioni congiunte degli Uffici di Presidenza e delle Conferenze dei Capigruppo della Camera e del Senato.

degli isolani, ossia gli abitanti delle isole, che si trovano sprovvisti del ciclo vaccinale completo o magari scelgono di non vaccinarsi e che nei mesi passati hanno avuto l'opportunità di circolare liberamente all'interno del territorio italiano.

il Ministero della salute aveva provveduto con l'emanazione di un'ordinanza, dando la possibilità di circolare all'interno delle isole minori ed escludendo le isole maggiori, quindi Sicilia e Sardegna. Nonostante vi sia stata una richiesta chiara, formale ed esplicita, anche attraverso gli organi di stampa, oltre che tramite i canali istituzionali, da parte del

La domanda che mi pongo rispetto a questa situazione è relativa ai danni che si determinano sul piano economico, a causa del mancato ingresso non solo dei residenti, ma anche

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle mille problematiche che attanagliano, oramai come una spirale asfissiante, la sanità regionale della Campania,

gennaio 2022, anche l'unico reparto di pediatria del presidio "S.S. Annunziata" del centro storico di Napoli, punto di riferimento per tantissime famiglie e i loro bambini, spesso appartenenti a fasce a fasce sociali meno abbienti e più in difficoltà. Ad esso afferivano pazienti provenienti soprattutto dal centro storico di Napoli e dalle periferie più difficili e disagiate della città, senza dimenticare tutti i Comuni dell'area metropolitana. Stante questa situazione, nell'attuale momento pandemico, come è possibile che in una città come Napoli, con circa un milione di abitanti e che, con tutta l'area metropolitana, arriva a circa 3 milioni di residenti, possa esistere, come punto di riferimento pediatrico immediatamente usufruibile per le emergenze e per l'assistenza, la sola struttura dell'ospedale "Santobono-Pausilipon", che, pur con tutte le sue competenze e professionalità, non può e non riesce a soddisfare tutte le necessità e le richieste dei piccoli pazienti, sia per il numero di accessi e di prestazioni richieste, sia per la sua localizzazione, non da tutti facilmente raggiungibile? Faccio appello al sindaco di Napoli, nella sua qualità di tutore della salute dei suoi concittadini, come previsto dalla legge n. 229 del 1999, ai direttori generali dell'azienda "Santobono-Pausilipon" e dell'ASL "Napoli 1" di Napoli di Napoli affinché facciano il massimo sforzo per trovare una soluzione rapida e immediatamente praticabile, che porti alle riaperture, in tempi strettissimi, del reparto di pediatria del presidio "S.S. Annunziata", inopinatamente chiuso. Rispondere alle emergenze pediatriche, alla richiesta di posti letto immediatamente disponibili, alla possibilità di accedere a un pronto soccorso pediatrico sempre attivo e prontamente accessibile è una necessità indifferibile, che fa parte della realtà quotidiana e non può attendere. Non può esistere, in un posto di primo soccorso, una guardia anestesiologica solo diurna e feriale, non considerando che le emergenze pediatriche possono verificarsi in qualsiasi momento. Vi sono situazioni, signor Presidente, di degrado, di povertà, di abbandono, che richiedono una pronta risposta, verso cui non si può restare indifferenti. In conclusione, signor Presidente, rinnovo l'invito agli amministratori a non aspettare che si verifichino situazioni irreparabili che coinvolgano i piccoli pazienti e gli stessi operatori sanitari, che prestano la loro opera con spirito di sacrificio e di abnegazione alla professione. Facciamo sì che il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione, e gli stessi diritti all'infanzia a ricevere un assistenza pediatrica adeguata non siano dimenticati o - peggio ancora - calpestati per la mancanza delle necessarie condizioni strutturali e organizzative. *(Applausi)*.